l'obbligo dell'accantonamento del Tfr durante il periodo di fruizione della cassa integrazione in deroga. gli onorevoli interroganti, con il presente atto parlamentare, chiedono al Ministero del lavoro di chiarire a quale soggetto spetti l'obbligo dell'accantonamento del trattamento di fine rapporto (TFR) durante il periodo dì fruizione della cassa integrazione guadagni (CIG) in deroga. ricordo che il TFR è un elemento della retribuzione il cui pagamento viene differito ad un momento successivo rispetto a quello relativo alla prestazione dell'attività lavorativa. Il TFR è costituito dalla somma degli accantonamenti annui di una quota della retribuzione rivalutata annualmente. In caso di fruizione del trattamento di cassa integrazione ordinaria o straordinaria, l'onere di accantonare le quote di TRF durante il periodo di sospensione rimane di norma a carico del datore di lavoro. Tuttavia, l'articolo 2 della legge n. 464 del 1972 prevedeva che in caso di licenziamento del lavoratore al termine del periodo di integrazione salariale, le aziende potevano chiedere all'INPS il rimborso del TFR limitatamente alla quota maturata durante il periodo ininterrotto di integrazione immediatamente precedente la risoluzione del rapporto. A seguito dell'abrogazione della legge 462 del 1972, operata dalla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 148 del 2015, il Ministero del lavoro ha precisato - con la circolare n. 24 del 5 ottobre 2015 - che le quote di trattamento di fine rapporto sono a carico del datore di lavoro. Rappresento, inoltre, che le quote di TFR relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro per stipula di contratto di solidarietà sono a carico dell'INPS, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati entro novanta giorni dal termine del trattamento di integrazione salariale. Per quanto concerne, invece, la fruizione del trattamento di cassa integrazione in deroga, il Ministero del lavoro ha precisato, mediante la circolare n. 4 del 2 febbraio scorso, che non possono essere rimborsate dall'INPS le quote di TFR maturate durante il periodo di sospensione dal lavoro per intervento del trattamento di integrazione salariale in deroga. la condizione di sospensione dal lavoro per intervento della CIG in deroga non rientra in alcuna fattispecie normativa che ne preveda l'indennizzo, essendo la relativa prestazione finanziata da risorse di natura non contributiva. Conseguentemente, la corresponsione delle quote di TFR maturate durante il periodo di intervento di integrazione salariale in deroga risulta a carico del datore di lavoro. che per i trattamenti erogati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 148 del 2015, anche nell'ipotesi in cui sopravvenga la risoluzione del rapporto di lavoro, dopo un periodo di CIG in deroga fruito dal lavoratore senza soluzione di continuità rispetto alla fine del periodo d'intervento di cassa integrazione salariale straordinaria, sono erogabili a carico della cassa integrazione guadagni solo

ringrazio molto il sottosegretario Bobba e mi dichiaro ampiamente soddisfatto della sua risposta. Credo infatti che la risposta del Ministero possa superare alcuni equivoci che in diversi territori del nostro Paese sono in corso tra chi sostiene che l'accantonamento del TFR sia dovuto dal datore di lavoro e chi invece ritiene che nulla sia dovuto dai datori di lavoro che si trovino in quelle condizioni.

mediante un proprio collaboratore, amici, conoscenti e parenti, hanno fatto sì che i due episodi siano stati immediatamente riferiti dal senatore Falanga alla presidente della Commissione antimafia, onorevole Bindi. Quest'ultima ha contattato il comandante generale dei carabinieri, che posto immediatamente il senatore Falanga in contatto con il generale di Napoli De Vita e con il colonnello comandante del gruppo con riferimento al territorio interessato (le ripeto, signor Presidente, che stiamo parlando del Comune di Torre Annunziata). Il senatore Falanga, nella sua esuberanza, in Commissione aveva sollecitato più volte un'indagine sull'amministrazione della città ed in particolare sulle ragioni di un mancato scioglimento del Comune, dopo che la commissione di accesso prefettizia - quindi l'organo *ad hoc* voluto dal prefetto affinché

il Governo li conosce e noi non riusciamo capire perché non si sia proceduto allo scioglimento del Consiglio comunale di Torre Annunziata. La commissione di accesso, la Commissione antimafia presieduta

di propria competenza il Ministero dell'interno intenda intraprendere al fine di far luce su questi fatti, di cui è stato destinatario un autorevole componente della Commissione di inchiesta sul fenomeno delle mafie.

Sono queste considerazioni, di grande preoccupazione, che hanno fatto sì che tutto il Gruppo firmasse questa interpellanza su questi atti intimidatori (ovviamente fatti propri anche dalla Commissione di inchiesta), che hanno visto un nostro autorevole collega, il senatore Ciro Falanga, vittima e ovviamente oggetto di questo attenzionamento. PRESIDENTE.

senatori, nel richiamare l'attenzione sugli esiti dell'accesso presso il Comune di Torre Annunziata effettuato dalla commissione di indagine nominata dal prefetto di Napoli per accertare eventuali infiltrazioni o condizionamenti di tipo mafioso, chiede di conoscere i motivi per i quali non si sia proceduto allo scioglimento dell'ente locale. Giova subito ricordare, in linea generale, che le conclusioni della commissione d'indagine non sono recepite acriticamente dal prefetto, al quale compete invece il potere e dovere di vagliarle, sentito anche il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio. Nel caso di specie il prefetto di Napoli, su conforme parere del predetto Comitato, ha ravvisato diverse criticità nella gestione dell'ente, ma ha ritenuto che non fossero tali da concretizzare i presupposti per lo scioglimento del Consiglio comunale, in quanto prive dei caratteri richiesti dalla normativa vigente sotto il profilo della concretezza, della univocità e della rilevanza. Nella valutazione l'autorità provinciale ha tenuto conto dell'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo secondo cui l'applicazione delle misure straordinarie va motivata con riferimento a risultanze obiettive circa la sussistenza dei collegamenti o delle forme di condizionamento. Rappresento, tuttavia, che, dopo il provvedimento con cui il Ministro dell'interno ha decretato la chiusura del procedimento, nel gennaio 2014 il prefetto ha invitato il sindaco di Torre Annunziata a porre in essere, entro il termine di sei mesi, le iniziative necessarie a rimuovere le forme di sviamento dell'attività amministrativa e gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico rilevati in sede ispettiva, che, ove persistenti, avrebbero potuto condurre allo scioglimento del Consiglio comunale per gravi violazioni di legge. Successivamente, la prefettura ha avviato nei confronti del Comune un attento monitoraggio che ha consentito di accertare l'avvenuta attivazione da parte dell'amministrazione locale di tutte le iniziative prescritte con l'invito-diffida, compresa quella più importante, consistente nello sgombero di Palazzo Fienga, ritenuto la roccaforte del sodalizio camorristico dei Gionta. Il prefetto ha comunicato che anche la procura della Repubblica e i vertici provinciali delle Forze dell'ordine hanno sottolineato il fattivo impegno profuso dal sindaco nell'opera di ripristino della legalità. Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto vengono richieste notizie anche sulle misure di protezione disposte a tutela dell'incolumità del senatore Ciro Falanga, componente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie, a seguito degli atti intimidatori consumati nei suoi confronti. gli onorevoli interpellanti fanno riferimento, come è stato ricordato, all'episodio verificatosi lo scorso 3 dicembre a Trecase, dove è stata incendiata l'autovettura dell'autista del senatore Falanga. L'incendio si è propagato anche all'autovettura parcheggiata dinanzi, che è risultata essere in uso al parlamentare, ma nella disponibilità dello stesso autista. Le indagini sull'episodio da parte del nucleo investigativo del gruppo carabinieri di Torre Annunziata e della procura della Repubblica competente sono tuttora in corso e coperte da segreto istruttorio. In relazione all'evento, il questore di Napoli ha disposto già dal giorno successivo la misura di vigilanza generica radiocollegata presso l'abitazione del senatore, intensificata anche in determinati orari. Nella riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia, convocata dal prefetto per il successivo 9 dicembre, il predetto dispositivo tutorio è stato ritenuto adeguato e, quindi, ratificato. Inoltre, è stato attivato un servizio di assidua vigilanza mobile presso tutti gli obiettivi dove è prevista la presenza del senatore, in particolare presso la predetta abitazione e in quella del suo autista.

Signor Presidente, l'interpellanza urgente che il Movimento 5 Stelle ha presentato il 28 gennaio scorso e di cui sono la prima firmataria nasce da un'altra risalente al mese di ottobre 2014 avente come oggetto lo stesso tema; anzi, per essere più precisi, lo stesso problema. Mi riferisco alla soppressione - prevista dal decreto *spending review* del 2012, esattamente dall'articolo 12, comma 20 del decreto-legge n. 95 - delle commissioni per l'abilitazione ad effettuare le attività connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali per il conseguimento del certificato di abilitazione alla manutenzione di ascensori Questo certificato fino al 2012 veniva rilasciato dal prefetto. Se con la prima interpellanza rilevavo un dato relativo al costo per il funzionamento della commissione in parola, che, stando alla Relazione sul rendiconto generale dello Stato del 2012 da parte della Corte dei conti, risulta assai modesto per lo Stato (circa 18.000 euro), evidenziando, inoltre, il grave danno che la sospensione degli esami sta procurando alle imprese operanti nel settore, le quali hanno investito hanno investito importanti risorse nella formazione del proprio personale, al fine di permettere ai tecnici, in particolare agli apprendisti, di acquisire le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per poter superare l'esame di abilitazione, con la seconda interpellanza riportavo un caso indirettamente connesso con la problematica in questione. Ed, invero, un articolo tratto dal quotidiano locale «Le iene sicule» del 23 gennaio 2016 riportava la notizia: «È finita soltanto con alcune lesioni e tanta paura:

Da un'altra fonte di stampa, risalente al mese di luglio 2015, si apprendeva la notizia di un'altra tragedia sfiorata; notizia riportata da un cittadino catanese coinvolto nella vicenda, che così ha dichiarato: «Prendiamo l'ascensore, ottavo piano, entrano altre persone, siamo in otto. All'improvviso una corsa velocissima, uno strappo, un contraccolpo orrendo: l'ascensore si blocca. Paura tanta, inizia a mancare l'ossigeno, siamo tanti, sei adulti, mio figlio di otto mesi e un bambino di otto anni circa. C'è pure una signora anziana. Gridiamo, nessuno ci sente. Il tempo scorre, suoniamo l'allarme, ma è afono: solo un debole cicalio. Non viene nessuno e io impreco, non capisco come una struttura pubblica che accoglie migliaia di persone non predisponga un servizio di sicurezza agli ascensori. Il mio piccolo piange senza soluzione di continuità e nessuno ci sente. I cellulari non hanno campo. Poi sentiamo delle voci: sono parenti e pazienti ricoverati, si prodigano, ma non ricevono risposte

È passata un'ora esatta, ci tirano fuori. Sono basito (...). Se quell'angelo custode non avesse sentito il pianto del mio piccolo Linus staremmo ancora lì, dentro l'ascensore, cianotici o svenuti». Come riportato dall'articolo di stampa, l'azienda ospedaliera Cannizzaro ha tenuto a precisare che l'evento accaduto il 18 luglio 2015 non è stato dovuto ad un cedimento, ma ad un blocco dell'ascensore, tanto che gli stessi vigili del fuoco intervenuti, nella loro relazione, l'hanno attestato quale presumibile causa del sinistro. L'ufficio tecnico dell'ospedale Cannizzaro pare che nell'immediatezza abbia scritto alla ditta, chiedendo le ragioni dell'accaduto e invitando a porre in atto ogni iniziativa utile a prevenire in futuro ulteriori analoghi guasti. Premesso che guasti del genere non dovrebbero nemmeno esistere o per lo meno dovrebbero essere evitati, non è inutile ricordare che, per eseguire in sicurezza le operazioni di manutenzione sugli ascensori, sono indispensabili competenze specifiche, conoscenze tecniche, teoriche e pratiche, nonché esperienza professionale. Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, rispondendo all'interrogazione 4-06728 del 4 novembre 2014, a prima firma dell'onorevole Crippa, ha evidenziato alcuni punti importanti fra i quali la necessità del certificato di abilitazione necessario per svolgere l'attività di manutenzione. Da qualche notizia pervenuta dal Ministero dello sviluppo economico risulta lo svolgimento di alcune riunioni, durante le quali sono state vagliate soluzioni per ovviare alla soppressione della commissione prefettizia, convenendo sull'opportunità di procedere ad una revisione della vigente normativa in materia di rilascio del titolo abilitativo. Il MISE ha comunicato alla sottoscritta che in data 8 aprile 2015 si è tenuta un'altra riunione, alla quale hanno partecipato alcuni rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Se durante la prima riunione il Ministero dell'interno ha sollevato la possibilità di riconsiderare la competenza prefettizia sulla materia, dalla seconda riunione - stando a quello comunicatomi è invece emersa la soluzione di ricostituire la commissione, rivedendone la composizione, al fine di prevedere esclusivamente rappresentanti dei Ministeri del lavoro e delle infrastrutture, incardinando tutto il procedimento, incluso il rilascio del patentino, in capo al Dicastero del lavoro che, oltre ad avere la competenza primaria, dispone di uffici periferici dislocati a livello provinciale. Sul punto, credo che la sua risposta potrà chiarire la posizione di questo Governo su un tema così delicato. Comprenderà bene che bloccare gli esami significa impedire il regolare svolgimento di procedure di assunzione nei casi di *turnover* in un comparto industriale come quello ascensoristico che francamente fino ad ora ha fatto vantare l'Italia non solo in Europa, ma anche nel mondo. Il timore che si cela e che abbiamo evidenziato senza troppi giri di parole nell'interpellanza di oggi è che vi sia una stretta connessione fra i fatti occorsi presso l'azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania e il blocco degli esami per conseguire il cosiddetto patentino, tale da lasciare il dubbio che dietro a questi casi si nascondano esempi di cattiva gestione o incauta manutenzione da parte di soggetti, possibilmente privi di adeguata preparazione tecnica; naturalmente vorrei venissero fugati. Attendo, quindi, di conoscere le valutazioni di merito, e di conoscere le concrete iniziative che il Governo intende intraprendere per risolvere definitivamente la situazione descritta. Concludo con le ultime notizie che apprendo da una associazione nazionale del settore, che comunica quanto segue: «Il MISE sta elaborando, da diversi mesi, uno schema di regolamento da approvarsi tramite decreto dei Presidente della Repubblica Repubblica n. 162 del 1999, la legge quadro sugli ascensori in Italia. Tale provvedimento è necessario per recepire nel nostro ordinamento la direttiva ascensori 2014/33/UE che, a partire dal 20 aprile 2016, dovrà sostituire la vigente direttiva ascensori 95/16/CE. Oltre al recepimento della direttiva, il Ministero intende apportare al decreto alcune modifiche di competenza nazionale, tra cui: la riaffermazione della competenza delle prefetture per il rilascio delle abilitazioni ai tecnici manutentori, aspetto fondamentale in quanto le relative commissioni prefettizie sono state soppresse e da oltre due anni non si tengono più sessioni di esame; la modifica dell'articolo 15 relativo alla manutenzione, precisando che il manutentore deve stilare un piano di manutenzione per ciascun impianto, su misura, in funzione delle sue caratteristiche e condizioni d'uso; modifiche minori agli articoli sulla messa in esercizio, verifiche e manovra di emergenza; l'introduzione dell'articolo 19*-bis*, rubricato «Adeguamento della sicurezza degli ascensori conformi alle norme vigenti fino alla prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile Mi chiedo se il Sottosegretario sia nelle condizioni di confermare quanto appena detto, ma soprattutto chiedo se il Ministero che oggi rappresenta è in grado di illustrarci le azioni adottate o adottabili d'intesa con la Regione Siciliana, al fine di appurare la reale applicazione della normativa vigente in materia. Vorrei ricordare che sulla sicurezza degli ascensori degli ospedali anche l'assessorato regionale alla salute dovrebbe mostrare attenzione. In ultimo, ritengo che questo Ministero debba assumersi l'onere di investire l'autorità giudiziaria del potere di indagine nel caso in cui dovessero emergere ipotesi di responsabilità in capo alla ditta autorizzata alla manutenzione degli ascensori dell'azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania, che, stando alle notizie a mia disposizione, non sarebbe una soltanto, o per lo meno magari a vincere l'appalto sono ditte che hanno nomi diversi, ma che di fatto hanno sede legale nello stesso indirizzo. Mi farebbe davvero piacere sapere se il Sottosegretario ha notizie specifiche su queste ditte, ma so bene che questa mia richiesta esula dall'oggetto dell'odierna interpellanza. Nulla di strano che potremo rivederci in un futuro prossimo per discutere di ditte vincitrici di gare d'appalto poco trasparenti

debbo dire molto dettagliata e ben documentata chiede al Governo quali iniziative intenda adottare al fine di superare lo stallo che si è venuto a creare nelle attività di rilascio dei certificati di abilitazione alla manutenzione degli ascensori, da quando i prefetti non possono più avvalersi, a tal fine, delle commissioni deputate ad esaminare la sussistenza dei requisiti tecnici necessari all'esercizio di quella professione. Voglio subito precisare che l'Amministrazione dell'interno condivide in pieno la preoccupazione per le difficoltà evidenziate dagli onorevoli interpellanti, tant'è che, al fine di prevenirle, ha consultato il Consiglio di Stato sull'esatta portata interpretativa della disposizione del decreto-legge n. 95 del 2012 soppressiva di tutta una serie di organismi collegiali operanti in regime di tra i quali proprio le commissioni in questione. In tale sede, l'Amministrazione ha sostenuto e argomentato l'infungibilità e la permanenza in vita di queste ultime, alla luce alla luce dell'assenza, all'interno delle prefetture, di professionalità tecniche in grado di assorbire le competenze demandate all'organo soppresso. Ricevuto dall'Alto consesso un parere di segno opposto a quello auspicato, questo Dicastero, unitamente alle amministrazioni rappresentate nella soppressa commissione, si è attivato per individuare il percorso più idoneo a ripristinare la funzionalità del settore a tutela dei profili di sicurezza e salute pubblica coinvolti e a soddisfacimento delle richieste occupazionali degli operatori del comparto. A tale scopo, si sono tenute varie riunioni interministeriali, nel corso delle quali si è anche ipotizzato - come evidenziato dagli onorevoli interpellanti - il trasferimento della competenza in materia ad altra amministrazione. Tale opzione non ha avuto seguito. D'altro canto, in linea con l'indicazione contenuta nel citato parere del Consiglio di Stato di fare ricorso a istituti disponibili nell'ordinamento a legislazione vigente, è stata presa in considerazione la possibilità di affidare le prove d'esame connesse al rilascio dell'abilitazione alla manutenzione degli ascensori a un organismo già presente nell'ambito delle prefetture: la conferenza provinciale permanente di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 189 del 2006. Tale ipotesi, però, si è rivelata inappropriata, essendo la conferenza un organo di supporto al prefetto nell'esercizio delle funzioni di coordinamento delle attività degli uffici periferici dello Stato e di garanzia del rispetto del principio di leale collaborazione tra questi ultimi e gli enti locali. Ulteriori perplessità si sono manifestate con riferimento all'ipotesi di avvalersi dell'istituto della conferenza di servizi di cui alla legge n. 241, che risulta orientato all'acquisizione di intese, concerti, nulla osta e atti di assenso nell'ambito di un procedimento amministrativo e, per questo, non si concilia

consista in un intervento normativo *ad hoc*, i cui dettagli sono in via di avanzata definizione in unità di intenti con la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli altri Dicasteri interessati. Come veicolo normativo è stato individuato il regolamento governativo di prossima emanazione, concernente la modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 per l'attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 33 del 26 febbraio 2014. Quanto ai contenuti della norma, è previsto lo svolgimento di una prova teorico-pratica innanzi a una commissione esaminatrice nominata dal prefetto territorialmente competente, composta da funzionari qualificati provenienti da diverse amministrazioni. All'esito positivo della prova, sarà il prefetto medesimo a rilasciare il certificato di abilitazione valido su tutto il territorio nazionale. Con riferimento all'ultimo quesito posto con l'interpellanza, il Ministero dell'interno si è attivato presso gli organi regionali preposti, che hanno fornito le seguenti informazioni. Premesso che gli ascensori delle aziende ospedaliere non rientrano nella categoria degli «ascensori in servizio pubblico» ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 9 marzo 2015, la conduzione degli impianti elevatori dell'azienda ospedaliera Cannizzaro è affidata ad apposita ditta, il cui personale addetto alla manutenzione è regolarmente abilitato ad espletare questo servizio ed effettua quotidianamente la verifica della funzionalità degli impianti stessi. A seguito dell'episodio ricordato di malfunzionamento verificatosi il 22 gennaio 2016, l'ascensore interessato è stato oggetto di ispezione e verifica da parte del servizio impiantistico e antinfortunistico dell'azienda sanitaria provinciale di Catania, che ha confermato che l'impianto ha funzionato in regime di sicurezza ed era stato oggetto di manutenzione periodica, programmata e straordinaria da parte della ditta affidataria del servizio, oltre che delle visite ispettive previste per legge. della salute ha approvato e autorizzato un progetto relativo alla sostituzione degli impianti elevatori dell'edificio "F" del polo ospedaliero Cannizzaro per un importo pari a circa 960.000 euro.

questo Parlamento ha bocciato anche i miei emendamenti. Nel frattempo, mentre i tavoli si riuniscono nelle sedi ministeriali, magari si poteva continuare a finanziare con 18.000 euro l'anno le commissioni prefettizie per evitare il *vulnus* legislativo. Vorrei ricordare che la Commissione europea, tra l'altro, con riferimento alla citata direttiva, ha rilevato un contrasto tra la normativa europea e la legislazione italiana rappresentata dal decreto ministeriale emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 11 gennaio 2010 e intitolato: «Norme relative all'esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone». Questo decreto ha solo una pecca: non si applica a tutte le tipologie di ascensori né a tutte le fattispecie di trasporto, perché in Italia il trasporto pubblico è ritenuto, evidentemente, Dovrebbe essere pacifico che la normativa nazionale non possa confliggere con quelle contenute nella medesima direttiva, la quale ha inteso garantire che gli ascensori, prodotti in qualsiasi Stato membro della Unione europea, possano liberamente circolare possano liberamente circolare negli altri Stati membri, senza venirne ostacolati dalla difformità dei requisiti tecnici diversi per essi. In proposito il decreto ministeriale dell'11 gennaio 2010, sopra menzionato, sottopone l'installazione e la messa in servizio della tipologia di ascensori, alla previa valutazione tecnica di un'apposita autorità interna: tale prescrizione duplicherebbe illegittimamente, ad avviso della Commissione, la procedura autorizzativa già disciplinata dalla direttiva al suo allegato II. Ammetto anche di non aver capito i motivi per cui da ventuno anni l'Europa aspetta che l'Italia si decida ad innalzare il livello di sicurezza dei suoi vecchi ascensori, soprattutto se teniamo conto che abbiamo impianti risalenti a prima del 1999, che non sono stati sottoposti a interventi di adeguamento e che, seppur siano manutenuti secondo la legge, sono pur sempre pericolosi. L'Italia ha, finora, disatteso l'invito ad innalzare il livello di sicurezza degli impianti preesistenti. Evidentemente, il Governo di allora era convinto di non dover mai invecchiare. La verità, signor Sottosegretario, è una sola e consiste nel fatto che questo Governo ha il dovere di adottare un atto a tutela della salute e sicurezza dei cittadini, nonché interventi di adeguamento volti a ridurre le probabilità di incidenti e infortuni. Auguriamoci che incidenti e infortuni non tocchino persone a noi vicine o noi personalmente perché, se il Movimento 5 Stelle dovesse scoprire che l'azione legislativa che volete intraprendere non è legata solo agli obblighi derivanti da quella raccomandazione,

senatori, con l'interrogazione all'ordine del giorno, il senatore Giarrusso, unitamente ad altri senatori, ha sottoposto all'attenzione del Governo l'attività di verificazione elettorale che la prefettura di Trapani è stata chiamata

Riguardo a tale adempimento, gli onorevoli interroganti hanno paventato che potessero esservi ritardi nell'esecuzione delle operazioni e che, quindi, la prefettura potesse avanzare una richiesta di proroga del termine fissato al 30 settembre 2014. Informo che l'attività di verificazione - disposta dal consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana con sentenza del giugno 2014 è iniziata il successivo 1° settembre. In merito alla tempistica della procedura seguita, va preliminarmente ricordato che la prefettura di Trapani,

i legali del sindaco eletto, unitamente a quelli del Comune di Alcamo, hanno comunicato la propria indisponibilità a presenziare alle operazioni programmate, giacché la data fissata ricadeva nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali. La prefettura ha pertanto ritenuto opportuno differire l'inizio della procedura al successivo 1° settembre non solo al fine di garantire il contraddittorio delle parti durante lo svolgimento La verificazione ha riguardato 35 sezioni elettorali su 41 e ha avuto ad oggetto, secondo le indicazioni fornite dal consiglio di giustizia amministrativa, una serie di schede elettorali connotate da particolari caratteristiche rientranti nelle tipologie indicate dallo stesso consiglio. Nel corso dell'attività di controllo è stata valutata, caso per caso, la sussistenza dell'elemento della riconoscibilità del voto, sulla base delle indicazioni contenute nella citata sentenza e degli orientamenti giurisprudenziali ivi richiamati. Segnalo che lo svolgimento dei lavori è stato connotato da notevoli difficoltà operative e ha richiesto un notevole impegno, sia per la considerevole mole di schede esaminate (per l'esattezza 22.307), sia per la situazione di accesa conflittualità tra le parti, assistite da numerosi legali, e le continue contestazioni, sovente rivolte anche al verificatore delegato dal prefetto di Trapani. Il procedimento di verificazione si è concluso il 18 settembre e la relazione dell'avvenuta verifica, unitamente a tutti gli atti connessi, è stata depositata presso la segreteria del consiglio di giustizia amministrativa il 29 settembre 2014, nel pieno rispetto del termine di esecuzione fissato, come detto, alla data del 30 settembre 2014, e dunque senza alcun ritardo. Sulla base della relazione, il consiglio di giustizia amministrativa, con decisione depositata il 19 marzo dello scorso anno, ha respinto nel merito la domanda di correzione elettorale proposta in primo grado, dando atto nella parte motiva che la verificazione si è «svolta in modo assolutamente ineccepibile e totalmente condivisibile». Per completezza, informo che il 6 giugno dello scorso anno il sindaco e la giunta municipale di Alcamo sono cessati dalla carica in conseguenza delle dimissioni rassegnate dal sindaco medesimo. Preso atto di ciò, il Presidente della Regione Siciliana, con proprio decreto del successivo 19 giugno, ha nominato un commissario straordinario per la gestione dell'ente fino alla prima tornata elettorale utile che si terrà nella primavera di quest'anno.

perché l'interrogazione faceva riferimento a tutto l'*iter* della vicenda esposta, che è stato caratterizzato da un diluirsi dei tempi, da ben due diverse decisioni della magistratura amministrativa di rigetto del ricorso - il che ha costretto a un terzo ricorso in revocazione solo dopo il rinvio a giudizio per voto di scambio per quelle medesime schede elettorali - e da un'ulteriore anomala lungaggine nelle attività della giustizia amministrativa, che - lo ricordiamo - sono attività in materia elettorale che richiedono procedure veloci,

verificazione. Lei ha detto bene, signor Sottosegretario: 22.000 schede di 35 sezioni esaminate all'interno del periodo di sospensione dei termini, che scade il 16 settembre. la richiesta di convocazione del 25 agosto è semplicemente un atto che mette una pezza all'interrogazione depositata il 22 luglio, quando noi abbiamo appreso che, subito dopo l'emanazione della comunicazione del provvedimento di verificazione alla prefettura, il funzionario delegato alla verificazione era semplicemente andato in ferie a luglio.

che hanno determinato le gravissime anomalie. Ricordiamo che c'è un procedimento penale per voto di scambio per le stesse schede che il consiglio di giustizia amministrativa ha ritenuto legittime e valide. Signor

Io ho personalmente esaminato i membri del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, che hanno deliberato il non scioglimento del Comune di Torre Annunziata.

mirata serie di quesiti inerenti alla sicurezza del lavoro nel predetto comando e, più in generale, nelle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. È un dato di fatto che il personale del settore operativo del Corpo nazionale, impegnato in operazioni di soccorso tecnico urgente per crolli o incendi, possa trovarsi esposto occasionalmente, per il breve periodo dell'intervento, a situazioni ambientali caratterizzate dalla presenza di fibre di amianto rilasciate in aria. In tali casi sono previsti mirati controlli sanitari, effettuati dal medico nei riguardi dei vigili del fuoco per i quali sia stata indagata, definita e notificata l'esposizione professionale, anche precedente, ad amianto sopra la concentrazione limite di 0,1 fibre per centimetro cubo d'aria. Si tratta di un importante intervento di prevenzione secondaria, che si aggiunge ai rigorosi interventi di prevenzione primaria, quali: l'abolizione dell'amianto, dove esistano materiali sostitutivi "sicuri"; il monitoraggio sistematico delle concentrazioni di fibre aerodisperse nelle aree ambientali "a rischio"; l'attuazione di procedure operative e tecniche idonee per evitare dispersioni incontrollate e inutili in tutte le operazioni che comportano interventi su materiali o strutture contenenti amianto. Ciò detto, passo ad illustrare le misure di carattere sanitario adottate nei confronti dei componenti delle due squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco di Macerata intervenuti nell'incendio da cui trae origine l'interrogazione. A seguito della segnalazione di sospetta esposizione ad amianto, effettuata da un capo squadra e confermata dal rapporto dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente Marche, i nominativi del personale intervenuto sono stati comunicati al medico competente, che ha attivato il protocollo sanitario concordato con la clinica di medicina del lavoro dell'ospedale regionale di Torrette di Ancona. In tale ambito, sono stati sottoposti alla prima fase di *screening* diagnostico quattordici vigili, quattro dei quali sono risultati positivi. Quindi il medico competente, tramite il comando provinciale, ha proposto a questi ultimi una TAC polmonare, al fine di disporre di una valutazione più approfondita dell'apparato respiratorio e dell'eventuale presenza di placche pleuriche. Egli ha proposto altresì, a tutti i vigili impiegati nell'intervento, la ripetizione dello *screening* con cadenza annuale. Inoltre, è stato disposto lo *screening* diagnostico per ulteriori 27 vigili, di cui 19 a scopo meramente cautelativo e 8 a seguito di un altro intervento di soccorso, per il quale il rapporto dell'ARPAM aveva rivelato la presenza di fibre di amianto nell'atmosfera. Pertanto, l'esigenza menzionata nell'interrogazione di effettuare uno *screening* cautelativo per almeno il 10 per cento del personale in servizio risulta soddisfatta, considerato che l'organico complessivo del comando di Macerata è di 180 unità operative. Con riferimento all'eventuale sussistenza nelle sedi di servizio del comando di Macerata di concause connesse alla potenziale esposizione ad amianto, ritengo doveroso far far presente, in linea generale, che la difesa della salute e della sicurezza dei vigili del fuoco costituisce una priorità assoluta dell'Amministrazione dell'interno; ragion per cui la presenza di materiali contenenti amianto nelle sedi di servizio del Corpo è stata oggetto di verifiche

è stata riscontrata l'assenza di componenti costruttive in amianto e ciò anche grazie all'attività di bonifica effettuata a suo tempo, in particolare presso la sede centrale ed il distaccamento di Civitanova Marche. Quanto, infine, ai dispositivi di protezione individuale utilizzati dai vigili del fuoco durante lo svolgimento delle operazioni di soccorso, assicuro che essi possiedono caratteristiche tecniche molto avanzate e garantiscono, quindi, *standard* di sicurezza e qualità spesso superiori superiori alle soglie previste dalle vigenti normative europee per la certificazione tipo. Soggiungo che, nelle ipotesi di rischi particolari, l'intervento operativo è affrontato con l'adozione contemporanea di diversi dispositivi in dotazione, in dotazione, a protezione sia del corpo che delle vie respiratorie. Presidente, mi dichiaro sufficientemente soddisfatto delle risposte che sono state fornite ai quesiti posti, non senza sottolineare l'esigenza di un costante monitoraggio della problematica per garantire la tutela della salute dei lavoratori che - come ha sottolineato il Sottosegretario - è indubbiamente un bene primario. Dico questo anche alla luce del fatto che in molte strutture industriali o produttive - parlo ovviamente anche del territorio del maceratese e della Regione Marche

gli stessi accertamenti sanitari, disposti dopo l'evento dell'ottobre 2014, evidenziarono la possibilità che le esposizioni fossero riconducibili anche a episodi precedenti e continuati,

la senatrice Ricchiuti pone all'attenzione del Ministro dell'interno la questione relativa alla posizione di 12 candidati che hanno partecipato alla procedura selettiva di stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari, bandita nel 2007, chiedendo in particolare iniziative volte alla loro riassunzione in servizio. Occorre premettere che i 12 candidati a cui fanno riferimento le interrogazioni hanno partecipato alla procedura di stabilizzazione, pur non essendo in possesso di uno dei requisiti di ammissione, in particolare quello di aver effettuato nel quinquennio precedente al bando almeno centoventi giorni di richiamo Inizialmente esclusi dal concorso, i predetti canditati, in virtù di una decisione cautelare del Consiglio di Stato, sono stati ammessi con riserva alle prove selettive. All'esito delle stesse, 11 di loro, essendosi collocati utilmente in graduatoria, sono stati assunti seppure con riserva dell'esito del giudizio di merito. Per un candidato non si è proceduto all'assunzione, in quanto convocato per l'assunzione, è risultato assente. Al riguardo, giova sottolineare che le assunzioni con riserva, come viene espressamente rappresentato dall'amministrazione agli interessati nelle lettere di convocazione, non determinano acquiescenza alle ragioni dei ricorrenti, ma rappresentano solo una mera esecuzione di ordinanze o sentenze di primo grado. Tant'è che nel caso in questione, a seguito del rigetto nel merito del ricorso da parte del Consiglio di Stato e su parere favorevole dell'Avvocatura generale dello Stato, l'amministrazione ha disposto l'annullamento della nomina a vigile del fuoco degli 11 interessati. Contro tale provvedimento questi ultimi hanno proposto ricorso rispettivamente al TAR Campania e al TAR Calabria, che, in via cautelare, hanno accolto la richiesta di sospensiva dell'efficacia del decreto ministeriale di annullamento della nomina La vicenda ha avuto ulteriori e più recenti sviluppi processuali. La posizione dei 7 ricorrenti al TAR Campania è stata definita con sentenza del 15 febbraio del 2014, che ha rigettato i ricorsi nel merito, ridando così efficacia al decreto di annullamento dell'assunzione degli interessati. Tale decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato il 22 dicembre 2014. Nella circostanza l'Alto consesso ha evidenziato come i rapporti di lavoro, sorti in via provvisoria in adempimento di un'ordinanza cautelare, non potevano indurre gli interessati a un legittimo affidamento circa la volontà dell'amministrazione di mantenerli in servizio, atteso che gli stessi non possedevano i requisiti per essere ammessi alla procedura di stabilizzazione. Per quanto concerne, invece, la posizione dei 4 ricorrenti al TAR Calabria, rappresento che gli stessi sono stati assunti con riserva presso il comando provinciale dei vigili del fuoco di Cosenza, nelle more della decisione di merito da parte del giudice amministrativo, il cui giudizio di primo grado risulta ancora pendente. Sulla scorta di quanto esposto, appare utile sottolineare come nella vicenda, in parte già definita e in parte in corso di definizione giudiziale, l'amministrazione non abbia alcun margine di discrezionalità. Essa, tuttavia, ha sempre manifestato considerazione per la difficile posizione dei soggetti interessati, come è dimostrato dall'adesione alle richieste di incontro formulate dai medesimi, i quali sono stati ricevuti allo scopo di fornire loro tutti i chiarimenti e le delucidazioni che le circostanze richiedevano.

Signor Presidente, il decreto ministeriale 18 aprile 2002, in linea con quanto previsto dall'articolo 930 del decreto legislativo n. 66 del 2010, in merito al transito di personale militare giudicato inidoneo al servizio militare incondizionato nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, prevede espressamente che il personale trasferito venga inquadrato nella qualifica corrispondente al grado rivestito al momento del trasferimento, secondo un'apposita tabella di equiparazione grado/area funzionale. La tabella compara i gradi di maresciallo ai profili professionali B3 (oggi seconda area "assistente"), ad eccezione del 1° maresciallo e del 1° maresciallo luogotenente, collocati in C1 (oggi terza area "funzionari"). Pertanto, gli infermieri militari che abbiano il grado di 1° maresciallo o di 1° maresciallo luogotenente transitano nella corrispondente terza area "funzionari" del ruolo dei dipendenti civili della Difesa. Il vigente ordinamento giuridico, altresì, prevede che il personale militare in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche può, a domanda, transitare nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa e di altre amministrazioni; tale facoltà è senza dubbio esercitabile anche dai militari infermieri. Di contro, il transito verso altre amministrazioni non è contemplato dal citato articolo 930 del decreto legislativo n. 66 del 2010, poiché lo stesso si occupa dei soli transiti di militari inidonei al servizio militare incondizionato. Nel dettaglio, per quanto riguarda il numero complessivo degli infermieri militari giudicati non idonei al servizio militare e transitati nei ruoli civili,

non sono passata dal servizio militare o dai corpi militari dei Ministeri. Il punto è capire se questi soggetti hanno la possibilità di avere un livello pari alla professione che esercitano, perché spesso mi sembra di evincere che vengono declassati rispetto al fatto che sono infermieri e, quindi, scendono di livello.

avere un'operatività maggiore e dare risposta a un'utenza molto più ampia, che non sia solo quella militare. In questo modo, invece, credo che l'offerta